colleghi, non appena l’emiciclo sarasgombrato da riunioni improprie si procedera con i lavori del pomeriggio.

L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonche´ ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonche´ di finanziamento delle opere per il G8

per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.200, 2.100 e 3.0.30. Esprime parere di semplice contrarietasulla proposta 1.0.250 (testo 2). Esprime parere non ostativo sulla proposta 3.3 (testo 2), con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che al capoverso 1-bis, dopo le parole: »20 milioni di euro« siano inserite le seguenti: »per l’anno 2008«; che al capoverso 1-ter le parole: »20 milioni di euro« siano sostituite dalle seguenti: »30 milioni di euro«. Esprime altresı parere non ostativo sulla proposta 3.5 (testo 3)».

2.100 Scarpa Bonazza Buora

votato. Nel confermare la nostra volonta di esprimere un voto favorevole, insieme ad una cinquantina di senatori (Viceconte, Bianconi, Gentile, Esposito, Morra, Contini, Carrara, Ghigo, Nessa, Mazzaracchio, Malan, Di Girolamo, Fazzone, Vetrella, Sarro, Compagna, Coronella, Giuliano, De Feo, Nespoli,

Non possiamo piu consentire che la situazione si protragga nel tempo, anche perche´ costa moltissimo alle casse dello Stato e degli enti locali; pertanto, soprattutto in un momento tanto difficile come l’attuale, e` necessario intervenire. Noi chiediamo che il Governo provveda a normare l’arbitrato

i fondi FAS per coprire ogni genere di intervento: e` una cosa indecorosa, della quale dovremmo vergognarci tutti.

lo scopriremo e lo denunceremo in quest’Aula, perche´ ha ragione chi ha detto che per gli arbitrati ci vuole una normativa di carattere generale. Debbo anche dire, signor Presidente, che era stata

vedete, dobbiamo fare chiarezza: non e possibile organizzare gli eventi con ordinanze, ce l’ha detto e raccomandato l’Unione europea, non una volta, ma cinque; pochi

a quanto previsto in tema di definizione agevolata delle disposizioni tributarie e contributive dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti conseguentemente al sisma del 1997 in Umbria e nelle Marche.

il tema del calcolo della compensazione da liquidare all’impresa appaltatrice da parte delle stazioni appaltanti per gli aumenti eccezionali dei prezzi subiti da alcuni materiali nel corso del 2008. dunque, lo scopo di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del nostro Paese e pesanti ricadute anche di ordine occupazionale.

alcuni emendamenti da noi proposti oggi relativi alle questioni legate al non obbligo di effettuare gare per la realizzazione delle opere pubbliche con lo scomputo di oneri. Non voglio recitarli ora ma voglio solo sottolineare la nostra parziale soddisfazione che in parte mitiga la delusione per non essere riusciti a portare avanti gli altri emendamenti. Capisco, peraltro, le ragioni che hanno portato il relatore ed il Governo ad esprimersi in maniera contraria, ma ribadisco il lavoro che abbiamo iniziato giada parecchio tempo rispetto all’assegnazione del 2 per cento per quanto riguarda le spese di progettazione. Da subito avevamo detto che, nell’attuale congiuntura economico-finanziaria, tale disposizione penalizzava fortemente i Comuni.

dei piccoli Comuni che, nell’attuale congiuntura, hanno estrema necessita di avere a disposizione tutti gli strumenti per poter amministrare nel migliore dei modi e nell’interesse dei cittadini di cui sono espressione. Pertanto, nonostante il piccolo rammarico

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, dico subito, per vostro e nostro reciproco sollievo, che depositeropoi il testo integrale del mio intervento perche´ sia

nonostante le significative novita intervenute nel corso dell’iter di approvazione, permane decisamente negativo e il nostro voto saraconseguentemente contrario. Cio nonostante, nel corso dei lavori in Commissione, e ancor piudurante i lavori in Aula, si sono registrati circostanze e interventi che non possiamo non cogliere e che, anzi, vogliamo sottolineare e segnalare alla vostra attenzione, anche e soprattutto a soprattutto a futura memoria. Mi riferisco, innanzitutto, alle risposte che il presidente Schifani ha voluto significare alle questioni poste dalla 5ª Commissione, per voce del suo onorevole Presidente e del past Presidente, collega Morando, tese a riportare il giusto ordine nella disciplina di approvazione degli atti, in occasione della sessione di bilancio. Ma piu in generale, mi riferisco anche agli impegni che la Presidenza ha assunto e sui quali ci attestiamo per il futuro, in ragione delle questioni

dei decreti-legge, che esulano perfino dalla questione specifica costituita dalla particolare situazione della sessione di bilancio, per investire direttamente l’ambito dei profili di costituzionalita, di corretto rapporto e di rispetto delle relazioni istituzionali. Purtroppo, nonostante i molti emendamenti ritirati, di cui vogliamo prendere atto, che avrebbero consentito di riportare il provvedimento nell’alveo della sua originaria impostazione e nel corretto profilo formale previsto dalle norme, il permanere di alcune significative eccezioni non puonon vedere il nostro piu convinto disappunto. E qui segnalo due questioni su tutte. il provvedimento consentiraad ANAS di incamerare i proventi derivanti dall’aumento del canone di concessione a carico dei concessionari, precedentemente finalizzato alle attivita di controllo e vigilanza sui predetti concessionari, indipendentemente dall’utilizzo per le finalita` di scopo. Lo consideriamo un atto grave, nel metodo assolutamente surrettizio ed estraneo all’oggetto del provvedimento, e nel merito in quanto consolida una prassi invalsa sui controlli e sulla vigilanza da parte di ANAS sulle concessionarie autostradali, che ediventata davvero insopportabile. Colleghi, e bene esser chiari: per noi la misura e` colma. Non solo assistiamo, com’estato denunciato in audizione di fronte al presidente di ANAS, il ruolo di interlocutore per conto dello Stato si limita a fare da passacarte, ma per giunta con quest’emendamento gli viene dato perfino il riconoscimento ed il compenso per la sua inattivita. Tanta grazia io credo davvero non la immaginasse neppure ANAS, che si era limitata ad accantonare le ingenti risorse non spese. E[]un atteggiamento che non possiamo tollerare specie quando non solo vediamo confuso il ruolo di chi deve essere controllato con quello di chi e chiamato a controllare, ma soprattutto quando non si appurano nemmeno le menzogne contenute nelle carte che attestano di riduzioni tariffarie sui sui pedaggi assolutamente inesistenti. Sorprende, al riguardo, che a dichiarazioni del tutto generiche ed evasive come quella di oggi riportata da Autostrade per l’Italia spa non segua una circostanziata precisazione dell’organismo preposto da ANAS al controllo e alla vigilanza,

a CAI, la futura compagnia aerea di riferimento, riteniamo che l’atteggiamento della maggioranza e del Governo sia stato sordo alle molteplici e garbate segnalazioni sia in Commissione che in Aula, finalizzate essenzialmente – e bene essere chiari – a circoscrivere la portata del provvedimento contenuto nella norma. Guardate, esemplicemente folle pensare di poter applicare la norma, che non consente l’automatica applicazione dell’articolo 2112 del codice civile per le grandi aziende in situazione di ristrutturazione economica e in amministrazione straordinaria, per altro con le pesanti modifiche gia intervenute recentemente sulla legge Marzano. Abbiamo chiesto e ci permettiamo, rivolgendoci direttamente al Governo, di continuare a chiedere una norma piuprecisa e piu puntuale che restringa e circoscriva almeno l’ambito di applicazione della norma approvata. Riteniamo che il Governo, nel suo stesso interesse, debba assumere un orientamento al riguardo, modificando – ci auguriamo – alla Camera il provvedimento, onde evitare effetti devastanti anche alla luce della crisi economica di rilevanti proporzioni che avvertiamo tutti incombere. Ci permettiamo di sollecitare questo intendimento anche a tempo scaduto, in forma sempre garbata, perche´ non eragionevole credere che il Governo intenda davvero insistere in questo proposito scellerato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione generale della societaitaliana e le sue dinamiche di natura economica e sociale impongono risposte alle aspettative generali poco compatibili con i tempi di carattere legislativo ordinario, cosı com’eper l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e i carburanti.

All’articolo 1 la compensazione prevista per l’aumento dei prezzi non eun ritorno alla revisione prezzi del passato ed e per questo che detta compensazione eoperata in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006. Il caso e quello dell’aumento di prezzi lamentato dall’industria delle costruzioni italiane e dai fornitori che hanno denunciato il rischio di fermo dei lavori ed i lavori minacciati da questo rischio sono quelli considerati vitali per lo sviluppo La difficoltadel nostro Paese di rispondere in maniera efficace alla realizzazione delle infrastrutture in pari agli altri Paesi europei rappresenta una delle ragioni di cio eproprio nel modo in cui legiferiamo, perche´ la norma cosı prevede, ma anche per la difficoltacon cui passiamo dalla progettazione alla realizzazione. Se almeno in parte queste difficolta debbono essere proprio intestate a qualcuno, questo non enella nostra parte politica, ma sicuramente in quella sinistra che ha voluto e difeso il diritto di veto di chiunque fosse contrario alla realizzazione delle opere, cosı come estato per tutte le piu importanti infrastrutture italiane negli ultimi anni, comprese quelle che faticosamente si stanno realizzando. Questa ela ragione per la quale, dovendo in specie rispondere ad impegni imperativi come il G8, si e utilizzato un provvedimento straordinario.

Per quanto riguarda la norma prevista per Alitalia, credo che essa sia veramente unica

n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (1175). La seduta e` tolta